osservare il principio di promozione delle pari opportunità non soltanto con riferimento all'articolo che ho sopra citato,

deve essere anche recepito e osservato in tutte le materie che si andranno a trattare e a toccare

Presidente, sono d'accordo anche perché abbiamo svolto un lungo lavoro in Commissione, che ha portato al recepimento di alcuni emendamenti da parte del relatore

«I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato».

nuova formulazione, più chiara e precisa, penso che ci possa essere una positiva considerazione da parte della maggioranza e del Governo sul fatto che i finanziamenti europei non possano essere sostitutivi. Quelli che nel quinto comma dell'articolo 119 vengono definiti come contributi speciali che lo Stato deve impegnare e devolvere per le situazioni di particolare disagio nella vita del Paese, devono essere comunque destinati e non essere, di fatto, sostituiti dai fondi europei. Questo è un principio che tutti quanti abbiamo sempre conclamato. Spero che il Senato, la maggioranza e il Governo vogliano

possano provocare delle situazioni di disparità e di ulteriore fuga, come già abbiamo visto, verso quei territori.

in considerazione positiva il metodo della programmazione pluriennale, l'attenzione ai territori montani, alle isole minori, alle aree sottoutilizzate del Paese e quindi mi sembra che con molta serenità e chiarezza

Passiamo alla votazione dell'articolo 24. BARBOLINI *(PD)*. Signor Presidente, sui principi che attengono al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livello di Governo si è discusso in Commissione e si sono introdotti dei criteri

tematiche che gli amministratori locali hanno spesso auspicato e cioè che ci sia non un generico, indistinto assembramento delle responsabilità, ma una verifica effettiva dei comportamenti che, se efficaci, orientati ad un pubblico servizio e a produrre benefìci per la comunità, possono anche consentire dei riscontri di premialità e rafforzare il principio e il valore dell'autonomia dei territori e delle amministrazioni. Per questo motivo, esprimeremo un voto favorevolesull'articolo 16.

per dare più elementi di ancoraggio e di riferimento nonché di evoluzione a tutto l'impianto delineato dal disegno di legge.

di spesa storica, modificandole in ragione dei costi standardsenza introdurre quell'elemento di coordinamento e di dinamicità nell'evoluzione del sistema che deve tendere a portare ad un livello di maggiore armonia armonia e corrispondenza ai fabbisogni definiti e individuati come obiettivi tutto il livello delle prestazioni che il sistema degli

Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 18.0.500, che per il Partito Democratico ha costituito uno dei punti fondamentali di tutta la discussione, lunga, complessa e io giudico positiva, che abbiamo svolto su questo disegno di legge.

l'assetto delle istituzioni, pur ritenendo che avrebbero dovuto essere prima definite le funzioni e gli assetti

Voglio tuttavia ribadire qui che questa è per noi una posizione abbastanza debole e di assoluta inadeguatezza rispetto al al quadro istituzionale di assetto delle autonomie locali che sarebbe necessario per una riforma del federalismo fiscale.

per il percorso politico che abbiamo iniziato; poi ci pronunceremo sui testi. Tuttavia rimane la nostra contrarietà di principio in quanto avremmo preferito e creduto necessario

che è una previsione costituzionale e che va in qualche modo prevista anche in questo testo, seppure in linea di massima. Non c'è una parola nel testo su tale

pur avendo con un nostro emendamento introdotto una norma per la partecipazione al fondo perequativo che sarà tutta da verificare secondo i loro Statuti, questo mio emendamento permetterebbe

far presente all'Aula è che stiamo parlando di norme transitorie, quindi anche l'80 e il 20 per cento vengono garantiti soltanto nella fase transitoria. Lo scenario finale

«Il Senato della Repubblica, esaminato il disegno di legge n. 1117, considerato il contenzioso tra Stato e Regioni prodottosi a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione e della relativa attuazione; rilevata l'esigenza di dare piena attuazione alle disposizioni costituzionali sull'attribuzione o il conferimento delle funzioni amministrative, impegna il Governo a promuovere, contestualmente alla predisposizione dei decreti legislativi, l'attuazione delle predette disposizioni costituzionali secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare con la sentenza n. 13 del 2004». PRESIDENTE. Invito il relatore

Signor Presidente, mi limito a fare una considerazione di carattere generale, che ovviamente riguarda la nostra proposta contenuta 20. La vicenda è nota e pertanto la ricordiamo solo in estrema sintesi. L'idea che il fondo perequativo per i Comuni sia gestito - non solo contabilmente, ma anche sostanzialmente dal punto di vista politico-istituzionale - dalle Regioni

Province, posto che veramente si sia deciso di mantenerle, di assolvere ad un ruolo paritario nel sistema istituzionale della Repubblica. Così è in base all'articolo 114 della Costituzione. E se così è - e abbiamo tutti accettato l'idea che tale norma costituzionale ha classificato come paritari i rapporti tra Stato, Regioni ed autonomie - non si può poi pensare che gli strumenti che la Costituzione attribuisce allo Stato per far crescere i Comuni

si reintroduce, peraltro, il principio dell'utilizzo della tassa patrimoniale e dunque dell'ICI, ancorché non per la prima abitazione, per tentare di far fronte alla copertura di funzioni degli enti locali, dei Comuni in modo particolare. È chiaro infatti che nel momento in cui si va verso un'attività di decentramento così ampia

espunta dal sistema di prelievo fiscale dei Comuni. Tutto ciò si tradurrà in un costo ulteriore per i cittadini a dispetto del principio tanto strombazzato, secondo cui il federalismo fiscale determinerà una riduzione dei costi

la conservazione dei sistemi museali o lo sviluppo dei sistemi di pubblica lettura. È altrettanto clamoroso che non si faccia cenno - nella situazione,

eliminare una limitazione che non avrebbe davvero ragione di esistere, risultando incomprensibile non solo per gli enti locali, ma anche per l'opinione pubblica nel suo complesso.

per il 19.504, su cui non ho avuto tempo di intervenire, l'osservazione è esattamente la stessa: la previsione di una delega concessa per un tempo illimitato contrasta con l'articolo 76 della Costituzione.

ma che è stato respinto sostenendo che a regime per i Comuni verrà definita la percentuale di partecipazione all'IRPEF. questo ragionamento può avere una sua coerenza; se però si prevede che ai Comuni debba essere assegnata una quota di partecipazione all'IRPEF, è bene definirne una percentuale nella fase transitoria.

riferimenti all'applicazione della legge del federalismo fiscale per poter dedurre i costi standard. Non si va a configurare una definizione delle funzioni fondamentali,

e con la discussione mi auguro addirittura che non vi sia neppure bisogno di quelle definizioni, che abbiamo trovato, puramente economiche e temporanee. Se, infatti, il Codice delle autonomie, risolti i due problemi principali, prenderà un'accelerata, potremmo non avere più neppure bisogno delle norme transitorie, credo a vantaggio di

voglio sottolineare che la scelta della senatrice Donaggio di collocare qui, nelle norme transitorie, una proposta di intervento per la determinazione, nella transizione fino all'applicazione a regime di questa legge, di una proposta di compartecipazione per i Comuni fissata una volta per tutte per l'IRPEF è una scelta, a mio giudizio, particolarmente avveduta. al senatore Azzollini - non hanno torto la maggioranza e il Governo quando, a fronte della richiesta di avere la determinazione di una compartecipazione fissa e quindi rendere dinamico il gettito per i Comuni nella soluzione a regime, in rapporto alla legge che stiamo approvando questa sia una scelta che si pone con una certa contraddittorietà rispetto ai principi generali, è vero che stiamo rapportandoci con i Comuni in modo assolutamente schizofrenico, cioè promettiamo loro una specie di mondo della felicità che verrà tra cinque o sei anni e, nel frattempo, c'è la dura realtà della scomparsa, per esempio, del gettito ICI, sostituito da trasferimenti che non compensano interamente il gettito stesso, c'è una realtà nella quale il Patto di stabilità vincola al di là di ogni ragionevolezza proprio i Comuni più virtuosi. Ecco perché, secondo me, non qui al Senato perché forse non siamo pronti, ma nella lettura della Camera sarebbe del tutto ragionevole che, anche per una interlocuzione positiva con il vasto movimento di sindaci che chiedono nell'immediato di introdurre una compartecipazione fissa all'IRPEF, nella transizione, cioè nelle norme transitorie, si provveda a dare una risposta. Se non nella misura del 20 per cento, in una percentuale più bassa in rapporto alla riduzione dei trasferimenti - si può discutere ma in via di principio credo che collocare nelle norme transitorie una proposta di compartecipazione fissa all'IRPEF durante la fase di transizione sia assolutamente razionale. Per queste ragioni mi rivolgo al Governo perché questa proposta venga presa in considerazione, come mi augurerei - naturalmente voterò a favore, assieme al mio Gruppo, di questo emendamento - almeno nella fase di discussione che seguirà. *(Applausi dal

Vorrei ricordare ai colleghi che, nel testo base, con riguardo alle funzioni del settore sociale era fatta eccezione per i servizi per l'infanzia e per i minori, per quanto riguarda appunto l'articolo di riferimento e le questioni ad esso attinenti. Abbiamo sollevato tale questione con molta forza e credo che questo sia un elemento molto importante, perché riguarda tutto ciò che i Comuni fanno per l'infanzia:

dai risultati finali e dagli atteggiamenti fermi ed intransigenti su tante questioni. Credo che sia un ottimo risultato su un settore molto sensibile e per questo il nostro voto sarà favorevole.

**Il Senato non approva.**

Presidente, credo di interpretare anche un parere favorevole del relatore e del Governo, dal momento che abbiamo lavorato fino a questa notte sui testi, sia noi che il Governo per

A me sono stati consegnati tre emendamenti due minuti fa, mentre lei stava per entrare in Aula. A conferma di quanto ha detto il senatore Astore, vorremmo avere il tempo di leggere questi emendamenti. Noi non abbiamo partecipato a nessun

delle norme statutarie che disciplinano il rapporto tra lo Stato e le Regioni autonome in materia di contribuzione per la realizzazione di opere pubbliche nei territori interessati.

peraltro con l'introduzione di un criterio che è funzionale non al riequilibrio economico e sociale dei territori ma solo a favorire i Comuni montani del Nord. Infatti, il criterio dell'adeguamento veloce al costo e al fabbisogno standard, così come disciplinato nell'articolo al comma 2, in italiano significa che per le politiche di coesione sociale, così come previste dal quinto comma preferiranno quegli enti e quei territori le cui amministrazioni si adegueranno velocemente al concetto di costo standard. È chiaro che tutto questo è inaccettabile e la nostra critica è radicale, e lo è ancora di più, signor Presidente, sull'emendamento 21.800, presentato presentato dal Governo, che propone di aggiungere alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 21, se il testo è confermato,

questa disposizione fosse complementare o aggiuntiva rispetto a quanto già vale per le Regioni a Statuto speciale, ma poiché non è così,

per determinare il contenuto di norme che sono costituzionali e per Costituzione riservate ad una fonte diversa. Lo stesso discorso riguarda anche la modifica che nel merito condividiamo, inerente i collegamenti con le isole minori.

ma un diritto: la continuità territoriale è garantita dalla Costituzione e non la si garantisce con i fondi speciali previsti dalla Costituzione per interventi che sono mirati solo ed esclusivamente a cercare di riequilibrare differenze territoriali. La continuità territoriale rientra nei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite sempre e comunque dallo Stato in via prioritaria. Di queste elemosine non sappiamo che farcene, questa è una ulteriore offesa anche all'intelligenza dei cittadini che vanno a votare.

caratteri locali di territori svantaggiati, nel primo caso, relativamente alle aree interessate dall'estrazione degli oli minerali, che producono un bene utile per l'intera collettività, e, nel secondo caso, per singole realtà territoriali svantaggiate.

per la parte che può essere ricondotta alla condizione di insularità e ai trasporti. Non sono d'accordo con le osservazioni che faceva il collega D'Alia

in una condizione di minor favore rispetto alle

positivo, contrariamente a quanto sostenuto dal collega D'Alia - di cui rispetto sempre le considerazioni, anche quando non le condivido - e certamente un grandissimo passo avanti in particolare per il Sud. È importante e fondamentale che, nel momento in cui si sceglie di considerare anche il deficit infrastrutturale come un elemento in base al quale effettuare la perequazione, conto naturalmente anche del disagio e delle difficoltà che vi sono in alcune aree del Paese, prevalentemente nel Sud, rispetto alla condizione di competitività cui il Paese stesso è chiamato, ancora di più, con il federalismo.

Ho ulteriormente riflettuto, anche rispetto alla deliberazione del Consiglio dei ministri,

qualche risorsa in più, l'unica oggettivamente rilevabile sia proprio la difficoltà conseguente al fatto di essere isole, quindi circondate dall'acqua.

realizzando così un lavoro che ha visto coinvolti i Gruppi politici ed il Governo nell'affrontare una questione importante per lo sviluppo del nostro Paese.

il presidente Vizzini ed il senatore Bianco. È un emendamento che si rivolge proprio alla particolare esigenza che la realtà insulare

parlamentare che all'epoca fu portato avanti dai Gruppi del centrosinistra. Credo pertanto che operare congiuntamente in questo disegno di legge, per scandire ancora di più l'esigenza di infrastrutturare e di servire meglio la realtà insulare, sia un fatto positivo. In Commissione la convergenza dei vari Gruppi ha prodotto l'emendamento 21.701; il Governo, da parte sua, in coerenza con iniziative annunciate in Consiglio dei Ministri e pubblicamente, ha voluto scandire in questa fase (dopo averlo detto, per la verità, anche in Commissione) un contributo importante. C'è da augurarsi che ora alle norme seguano i fatti. Il vero problema è infatti realizzare, soprattutto nella realtà della Sardegna e altrove, quelle infrastrutture di cui si avverte una storica, ma anche urgente necessità. Voteremo quindi con convinzione a favore del testo che scaturirà

una leggera deviazione da una prassi parlamentare consolidata. Siamo in presenza di un emendamento di iniziativa parlamentare (a prima firma non di un senatore del Partito Democratico, ma di un senatore del Popolo della Libertà), che conteneva delle norme sulla continuità territoriale di alcune aree del nostro Paese. Tale emendamento ha ha parlamentarmente un diritto di primogenitura, a mio parere. Su di esso è intervenuta un'iniziativa del Governo, che ha colto non solo il senso, ma anche la lettera dell'emendamento 21.701 e vi ha apportato quelle che io giudico delle limitate modifiche. Oggi noi mettiamo in votazione l'emendamento del Governo e non mettiamo in votazione, mi sembra, l'altro emendamento.

Governo e Parlamento. Credo che sarebbe stato meglio se il Governo avesse chiesto ai presentatori di riformulare l'emendamento da loro presentato, lasciando che solo

dinanzi alla disponibilità del presidente Vizzini, concessa dal Governo, di riformulare il proprio emendamento in modo identico a quello del Governo, del Governo, si arriverebbe, presidente Zanda, alla votazione di due emendamenti identici, quello del Governo e quello del presidente Vizzini, con l'accoglimento del subemendamento del senatore Cabras.

ma premia l'iniziativa parlamentare, alla quale questa Presidenza non può che essere sensibile naturalmente, dovendo tutelare anche le iniziative dei singoli parlamentari, a maggior e dal presidente Pistorio; quindi da parlamentari che hanno seguito da vicino, in 1a Commissione permanente, il tema del federalismo fiscale. Questa è la sintesi. Vediamo pertanto se possiamo muoverci in questo solco durante l'espressione dei pareri e le votazioni.

di contenere i guasti di una intrusione nelle prerogative autonomistiche ma vorrei senza polemica dire al collega Cabras che

così non ci giriamo attorno ed evitiamo il conformismo del «volemose bene» anche quando sul merito ci sono divisioni profonde come in questo caso - per cui tutti gli organi di programmazione economica, dal CIPE in poi, nella fase transitoria del federalismo fiscale, vengono sostituiti da una cabina di regia composta da quattro Ministri, che devono fare la ricognizione delle opere pubbliche e degli interventi mirati all'attuazione del quinto comma dell'articolo 119, sul piano politico è legittimo, purché ne siamo consapevoli, ma per noi non va bene. In secondo luogo, se questa disposizione fosse aggiuntiva al rispetto, perché vi è la clausola costituzionale che le condizioni di maggior favore sotto il profilo dell'autonomia si attribuiscono anche alle Regioni a Statuto speciale, allora saremmo d'accordo. Ma poiché il testo, così come scritto, sembra essere sostitutivo delle norme statutarie che prevedono come lo Stato intervenga anche nelle materie, di cui per garantire la coesione sociale, vi renderete conto che questo determina che i fondi che lo Stato dovrebbe dare alle Regioni a Statuto speciale, da anni ed in particolar modo - parlo per la Sicilia - sul contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto, ce li scordiamo e ci scordiamo il contenzioso in atto, che serve a regolare in maniera certa e stabile i rapporti finanziari, federali, quelli sì veramente federali, tra lo Stato ed il sistema delle autonomie speciali.

ripartizione delle risorse, anche con riguardo al criterio della insularità e per garantire diritti costituzionalmente garantiti, come

vanificate esattamente il sistema attraverso cui lo Stato deve continuare ad intervenire in via ordinaria per garantire alcuni diritti costituzionalmente garantiti per i territori più svantaggiati. Questo è il tema politico. Dopodiché, rispetto le opinioni di tutti, ma almeno cerchiamo di stare alle questioni così come sono scritte nelle norme che si stanno votando.

influisce sull'assetto generale, porti una nuova indicazione su un tema importantissimo, quello dell'energia. la valutazione della capacità produttiva energetica reale e potenziale di ciascuna Regione sia oggi importante, soprattutto perché ciò ci consente di ricollegarci con gli articoli successivi. Alcune Regioni pagano infatti un prezzo più alto;

voteremo a favore dell'articolo 21 perché, come ho detto illustrando il mio emendamento, si tratta di un significativo passo avanti: viene sancito il principio che la perequazione non può non tener conto anche della condizione infrastrutturale in cui versano le differenti Regioni del Paese. Alla preoccupazione avanzata dal collega D'Alia, che ha formulato l'emendamento soppressivo, vorrei timidamente che l'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana è norma costituzionale e non può essere modificato da una legge ordinaria. È elementare che sia così ed egli lo sa perfettamente.

nell'articolo 24 affrontiamo il tema delle Regioni a Statuto speciale. Più volte abbiamo richiamato la necessità, da un lato, di garantire la la specificità e il carattere pattizio del rapporto che si ha con queste Regioni e, dall'altro, c'è stata sempre la preoccupazione di evitare che la specialità paradossalmente nel riassetto federale potesse essere un limite o comportasse meno opportunità. Ecco perché con questo articolo si tenta, invece, di conciliare le due dimensioni:

abbiamo dovuto inserire, a mio avviso giustamente e alla luce anche del dibattito che qui si è svolto, la necessità di una perequazione infrastrutturale. Quindi, si ritiene che la perequazione infrastrutturale è comunque un elemento che deve svolgere una sua funzione. Gli emendamenti 24.502 e 24.504 che ho presentato vanno in questa direzione nella parte che

alle dotazioni infrastrutturali e ai servizi sociali e sanitari. Inoltre, signor Presidente, un aspetto particolare

consentire a queste Regioni di passare da una specialità tutta giocata sul piano della rivendicazione storica ad una specialità che, invece, investa con coraggio sul piano della progettualità, della capacità di cambiamento, di competizione, di innovazione che le Regioni a Statuto speciale, soprattutto la Sicilia e la Sardegna, devono essere

l'emendamento 24.506 indica la necessità di definire in modo pattizio la piena attuazione delle norme per le Regioni a Statuto speciale che nei loro Statuti prevedano condizioni di maggiore vantaggio nell'accertamento e riscossione dei redditi delle imprese che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, in modo tale che nell'accertamento dei redditi venga determinata la quota da attribuire agli stabilimenti ed agli impianti medesimi. È una vecchia questione, mai risolta definitivamente, che nel che nel contesto attuale del riassetto federale e del ruolo delle Regioni a Statuto speciale ritengo debba finalmente trovare una strada

grazie.

tutte le disposizioni che enfatizzino la specialità; tale enfatizzazione si configura, infatti, come una sorta di sottrazione agli obblighi del quadro della solidarietà nazionale.

una verifica da parte del Parlamento dei risultati della negoziazione tra il Governo nazionale e quelli regionali nella fase di stesura delle norme di attuazione degli Statuti, ritiro l'emendamento.

che qualunque voto aggiuntivo non legittimato dalla presenza del senatore è veramente superfluo ai fini politico-parlamentari, al di là del malcostume insisto in sé. Metto

dei costi della politica, a migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini e a rendere più efficienti i rapporti tra cittadini e istituzioni.

(norme di salvaguardia e garanzia, su cui abbiamo molto insistito nel lavoro di Commissione), e cioè che durante tutta la fase transitoria si abbia attenzione a monitorare l'andamento dei costi e delle spese, in modo da evitare appesantimenti della pressione fiscale.

a tenere sotto controllo - auspicabilmente, perché questo è il senso e la finalizzazione di tale intervento sulla spesa pubblica - e ad avere un processo di graduale abbassamento e riduzione della pressione fiscale complessiva.

ove si realizzino questi obiettivi, la priorità del beneficio sia riconducibile primariamente ad alcune tipologie di cittadini, in particolare alle figure dei lavoratori dipendenti a basso reddito e dei lavoratori precari e discontinui; alle famiglie con figli minori e pensionati a basso reddito; all'attività di sostegno ed accompagnamento della ricerca e dell'innovazione delle piccole e medie imprese, data la rilevanza che questo

attuare questa politica lo fa intervenendo sulle sue basi imponibili e non, come abbiamo tristemente conosciuto nell'anno in corso, andando a pescare sulle basi imponibili di altri soggetti, come è avvenuto con l'ICI, determinando tutte le conseguenze negative di cui i Comuni si lamentano nell'esercizio della loro attività ordinaria. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'emendamento 25.701 riguarda l'articolo 25 del disegno di legge, che è la cerniera economico-finanziaria dell'intero provvedimento.

tant'è vero che al comma 1 questo articolo stabilisce un paletto importantissimo e cioè che nell'attuazione del federalismo fiscale si dovranno rispettare tutte le condizioni del patto di stabilità con l'Unione europea. È questa una prima garanzia che l'attuazione del provvedimento al nostro esame non determini sfondamenti negli equilibri finanziari del Paese. Tuttavia, signor Presidente, mantenere il patto di stabilità con l'Unione europea significa garantire i saldi di bilancio, non l'andamento del totale della spesa e del totale delle entrate fiscali. È evidente che un saldo di bilancio può essere ottenuto aumentando la spesa e il prelievo fiscale.

fondamentale per un patto chiaro che il federalismo deve rappresentare come strumento strategico di politica economica, di democrazia, di maggior potere dei cittadini e di minor potere degli apparati pubblici a qualunque livello essi facciano riferimento: Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane. Pertanto, signor Presidente, dobbiamo smascherare una profonda ipocrisia, perché per due mesi ci è stata chiesta in Commissione la disponibilità dei dati e delle simulazioni. Ebbene, il lavoro proficuo e serio svolto in Commissione ha condotto a capire una cosa fondamentale: ad oggi i dati sono stati resi disponibili da due mesi ai membri della Commissione - e quindi a quest'Aula del Senato attraverso le audizioni che abbiamo svolto con tutti gli organi competenti che producono queste informazioni. Diverso è l'argomento con il quale si chiedeva, e si chiede tuttora, di svolgere le simulazioni per capire come l'applicazione del federalismo fiscale inciderà nella ripartizione e allocazione delle risorse tra i vari livelli di governo e i vari territori. Ebbene, tali simulazioni, come correttamente

un provvedimento ampiamente condiviso con il relatore di maggioranza e il relatore di minoranza.

morbido, graduale e ragionevole. Infatti, l'emendamento dice che nei primi due anni verrà attuato il federalismo, nei due anni successivi

nei tre anni successivi questo tetto dovrà scendere al 40 per cento. Ebbene, ci vorranno sette anni, signor Presidente, per ritornare alla pressione fiscale

non per tagliare il deficit pubblico - perché sappiamo che il deficit pubblico del 2008 è superiore a quello del 2006 - bensì per consentire uno sperpero ulteriore della spesa pubblica. Allora, giù la maschera dell'ipocrisia! Se siamo d'accordo sul rigore finanziario occorre porre il vincolo europeo sul saldo, ma anche prevedere un percorso ragionevole, morbido, lungo nel tempo per poter dire che, almeno tra sette anni, torneremo a pagare le stesse tasse che, in totale, i cittadini italiani hanno pagato nel 2006,

strumento di democrazia, di equa ripartizione delle risorse, di responsabilità tra entrate e spese di tutti gli enti che governano il Paese, e dunque di responsabilità verso i cittadini. Infatti, è giusto dire ad ogni cittadino, ad ognuno di noi, quanto deve pagare al Comune e per che cosa, quanto alla Provincia e per che cosa,

Colleghi, vi prego, siamo ormai al termine, a pochi minuti dalla conclusione della seduta e spero anche dall'esame le trasmetto il testo dell'ordine del giorno, che prego un assistente di portarle. Le chiedo di leggerlo e su questo chiedo il voto elettronico

o qualcuno in quest'Aula è in grado di offrire al senatore Baldassarri gli elementi di fatto in base ai quali un emendamento come quello può essere ritirato, ma ieri il ministro Tremonti ci ha detto che non è in grado di farlo, oppure una norma di chiusura e di salvaguardia è più che necessaria e non si capisce come sia possibile chiederne il ritiro. l'articolo in oggetto dispone le norme di salvaguardia sia in relazione al rispetto del patto di stabilità e crescita, sia in relazione alla pressione fiscale. È auspicio di tutti e credo sia da tutti condiviso che si potrà arrivare ad una riduzione dei costi e quindi ad una riduzione della pressione fiscale e mi auguro anche ad un miglioramento dei servizi. Ritengo che

Presidente, le chiedo di poter conoscere il testo dell'ordine del giorno (ormai l'emendamento, per decisione del suo proponente,

un testo che traduce letteralmente il contenuto dell'emendamento. Quanto sto per dire vale per l'emendamento, così come per l'ordine del giorno di conseguenza. Avrei votato contro questo emendamento, e voterò personalmente - al di là dell'orientamento del mio Gruppo, che non conosco - anche contro l'ordine del giorno, a meno che a meno che (e questo sarebbe valso per l'emendamento, esattamente come vale per l'ordine del giorno) il proponente non sia disponibile ad introdurvi un punto, che considero assolutamente essenziale in questo confronto, e la cui assenza mi fa ritenere che l'emendamento (e il conseguente ordine del giorno) sia solo un'operazione di tipo propagandistico. Perché in Italia abbiamo una pressione fiscale così elevata? Se non rispondiamo con precisione a questa domanda, tutto il dibattito conseguente è privo del necessario fondamento. La risposta la conosciamo tutti:

degli altri grandi Paesi dell'Unione europea, perché abbiamo un elevato livello del debito pubblico accumulato nel corso degli anni e perché, malgrado gli anni passino, non siamo stati in grado - né il centrosinistra, diciamo le cose come stanno, né il centrodestra - di mettere davvero e definitivamente sotto controllo l'evoluzione della spesa corrente primaria.

spero che presto tornerà al Governo il centrosinistra, per cui, se non ci avrà pensato il centrodestra, dovremo pensarci noi. Ma il punto cruciale è che si può credibilmente affrontare il tema della definizione anno per anno, e pluriennalmente, di un obiettivo di pressione fiscale in riduzione (sapete che la pressione fiscale è la somma di tutti i tributi e contributi in rapporto al prodotto interno lordo), soltanto se contestualmente ecco quello che non c'è - nel Documento di programmazione economico-finanziaria, e nella relativa risoluzione parlamentare, è contenuto un obiettivo separato, ed altrettanto individuato puntualmente, di riduzione della spesa corrente primaria. In tutti gli altri casi la definizione di un obiettivo di riduzione della pressione fiscale è priva del necessario fondamento nella realtà della scelta politica di gestione di bilancio. Ecco perché, se il senatore Baldassarri introduce nell'ordine del giorno così come non ha fatto invece nell'emendamento - l'esigenza che nel DPEF, come qui è scritto, ci sia, certo, un obiettivo di riduzione della pressione fiscale e contemporaneamente un altrettanto puntuale e impegnativo obiettivo di riduzione della spesa corrente primaria, allora abbiamo un orientamento convergente e possiamo votare assieme. Al contrario, se non c'è l'obiettivo di riduzione della spesa corrente primaria, si tratta di una presa in giro e onestamente, professor Baldassarri, questo non è il posto, per quanto mi riguarda.

le maggiori risorse finanziarie rese disponibili a seguito della riduzione delle spese determinino una riduzione della pressione fiscale dei diversi livelli di governo». Ed è chiaro che qui è incluso il discorso della spesa corrente.

del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria».

con l'ordine del giorno del professor Baldassarri, trova una chiusura che mi pare soddisfacente. Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1117 e connessi

considerato che: l'attuazione del decentramento fiscale e dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali costituisce una riforma strutturale dell'ordinamento fiscale e finanziario della Repubblica; la pressione fiscale complessiva riferita all'anno 2006 è stata del 40,6 per cento in rapporto al PIL e nel 2008 tale percentuale è salita fino al 43,3

e quindi l'imponente aumento della pressione fiscale è stato sostanzialmente inutile ai fini del contenimento di tale rapporto *deficit*/PIL, essendo stato utilizzato per ulteriori aumenti della spesa pubblica; l'obiettivo finale dell'introduzione del federalismo fiscale consiste nel miglioramento della qualità della spesa pubblica, nel suo contenimento e nella riduzione della pressione fiscale complessiva, impegna il Governo a fissare il limite di pressione fiscale complessiva dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL nel Documento di programmazione economico-finanziaria, in modo tale che dall'attuazione della presente legge e, comunque, dall'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della stessa, sia assicurato il rispetto di tale limite e definito di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo; a fissare entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva ad un livello non superiore al 42 entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente a un livello non superiore al 40 per cento; e a fissare quindi, successivamente a tale termine, tale percentuale a un livello non superiore a quello della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno, impegna altresì il Governo, nel pieno rispetto dei vincoli concordati in sede comunitaria al fine di garantire il percorso di rientro del rapporto *deficit/*PIL fino al suo completo completo azzeramento, a proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente e senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva. A tali fini entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

a specificare meglio l'ultimo comma dell'ordine del giorno, introducendo, dopo le parole «a proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente»

che il senatore Morando aveva richiesto, ma che corrisponde, dato il testo, a quello che volevo esprimere sia nell'ordine del giorno sia nell'emendamento. Ringrazio il rappresentante per aver accolto questo impegno politico, fondamentale ai fini di questo provvedimento. Per la verità, ritengo che il testo dell'ordine nel giorno accolga in parte quanto da me richiesto, ma non accolga il punto fondamentale. Propongo al senatore Baldassarri - che immagino possa concordare, quindi lo faccio veramente a fini di

«a fissare nel Documento di programmazione economico-finanziaria un preciso e distinto obiettivo di spesa corrente, di spesa corrente primaria, di spesa in conto capitale dello Stato centrale e di ogni comparto della pubblica amministrazione». Se c'è l'introduzione di questa precisa frase, allora è quello che ho sostenuto. Se invece abbiamo la determinazione puntuale di un obiettivo di pressione fiscale, addirittura con una percentuale e la sede - il DPEF - nella quale viene individuato quell'obiettivo, e poi abbiamo un fervorino sulla riduzione della spesa corrente primaria, allora non sono d'accordo e non voto a favore dell'ordine del giorno.

Ministro Calderoli, è arrivato in questo momento un nuovo emendamento, il 21.0.100 del relatore, sulle norme transitorie per le Città metropolitane, che sostituisce